Grazie, indicano un'incidenza addirittura sui meccanismi democratici e sul funzionamento delle istituzioni da parte di coloro che effettuano detti accessi, attività spionistiche e di intrusione nella vita altrui, peraltro in un ambito ampiamente e specificamente protetto dalla Costituzione. Auspico Auspico - immaginando che questo sia - che tutte le forze politiche qui rappresentate si rendano disponibili, a cominciare naturalmente da quella che io ho l'onore di presiedere qui, per ogni attività che possa essere utile a fare chiarezza su questi fenomeni e, eventualmente, a prendere iniziative legislative per contrastarli e prevenirli. *(Applausi)*.

grave e allucinante sotto molti aspetti, che riguarda dati rubati, *privacy* violata, spionaggio industriale

solidarietà che estendiamo, colleghe e colleghi della maggioranza, a tutte le italiane e gli italiani che si trovano nella stessa condizione della famiglia del presidente La Russa. Russa. Se c'è un problema grande che la società digitale ci chiede di affrontare, questo è il problema della *privacy*. Dobbiamo avere chiaro, presidente Malan, che *privacy* non significa nascondere agli altri la vita privata, ma evitare che la vita privata degli altri irrompa dentro quella di ognuno di noi. Su quello che è successo a Milano, signor signor Presidente, non c'è ancora stata una parola del Governo, che sia una. Il Paese da tre giorni prova a chiedersi che cosa sia successo dentro gli apparati dello Stato e dentro i nostri sistemi di sicurezza, ma dal Governo non è arrivata alcuna parola. Vogliamo sapere, signor Presidente, che cosa pensa il Governo, e per questo abbiamo chiesto che la Presidente del Consiglio e i Ministri competenti vengano in Aula a riferire. Non è sufficiente dire che i colpevoli verranno puniti, perché in questo caso è evidente che c'è un serissimo problema connesso alla sicurezza non solo interna, ma anche di molte banche dati sensibili. Dalle notizie che si evincono, è una vicenda di *dossier* predisposti nell'interesse di autorevoli esponenti politici contro altri esponenti politici, tutti purtroppo rigorosamente di destra. E mi riferisco ai committenti. Allora, signor Presidente, chiediamo alla maggioranza di unirsi a noi nella richiesta di dimissioni di

sistema l'istituto dell'autosospensione, quando si è al vertice di un'azienda o di un ente pubblico, men che meno di una fondazione. Ci auguriamo che la destra tutta unita, a partire da quella milanese che fa finta di non capire cosa sta succedendo - si unisca a noi non solo nella richiesta di dimissioni di Pazzali e di coloro che, come lui, ricoprono ruoli pubblici, ma anche nella richiesta di chiarimenti da parte del Governo, a partire dalla Presidente del Consiglio. Sono convinto che, se uniamo le forze, facciamo chiarezza su questa vicenda e difendiamo insieme non solo la credibilità delle istituzioni repubblicane, ma anche il funzionamento degli apparati dello Stato, che è evidente che sono stati a dir poco vulnerati. *(Applausi)*. PRESIDENTE.

signor Presidente. Le vicende e le notizie che ci stanno arrivando da Milano sono estremamente preoccupanti. Dal nostro punto di vista, il Parlamento e le istituzioni, nel pieno rispetto delle competenze, degli equilibri dei poteri e delle garanzie attribuiti ad ogni livello istituzionale, debbono fornire risposte adeguate in tempi rapidi. Signor Presidente, stiamo parlando di un dossieraggio che ha riguardato - così narrano le cronache più di 800.000 *file*. È come se l'intera città di Torino fosse stata illegalmente dossierata. dossierata. Pare che addirittura il *server* del Quirinale sia stato bucato. Certamente è stata coinvolta la Camera nella quale siamo seduti, perché il Presidente del Senato, al quale va la nostra solidarietà, insieme con la sua famiglia, è stato oggetto di un illecito esercizio di dossieraggio. Certamente riguarda questa Camera, perché un ex Presidente del Consiglio che siede qui ed ed è *leader* di uno dei partiti dell'opposizione, il senatore Matteo Renzi, è stato oggetto illegale di dossieraggio. Questi aspetti di per sé già meriterebbero un'adeguata risposta, non in funzione di generiche garanzie, ma della tutela degli equilibri democratici del Paese. i pubblici ministeri di Milano hanno usato frasi di fuoco e hanno parlato di eversione. Sin qui potremmo dire che sia una valutazione di parte, perché occorrerà capire cosa decideranno gli altri giudici, ma il Presidente del Consiglio, nei giorni scorsi, ha usato la stessa parola utilizzata dai pubblici ministeri di Milano: ha parlato di eversione, ha detto che siamo vicini all'eversione. Se le cose stanno in questi termini, noi pensiamo che il Parlamento debba dare immediata risposta, quantomeno su tre livelli. Il primo livello livello riguarda le competenze di ciascuna responsabilità interna e ci risulta che già il Copasir e la Commissione antimafia stiano lavorando su questo versante, ma ciò non è sufficiente e di per sé non è esaustivo. Noi crediamo che sia indispensabile un'informativa immediata della Presidente del Consiglio, che deve venire in quest'Aula a riferire in dettaglio delle questioni, anche perché gli squarci che arrivano dalla vicenda

o sia stato intercettato, o se questa malevola attività sia frutto di corpi infedeli all'interno delle strutture della Repubblica. Non lo sappiamo, ma certamente già solo questi sono inquietanti interrogativi che devono essere immediatamente chiariti in questa sede da parte del Governo. Riteniamo anche, per la gravità dei fatti, per il fatto che sia stato coinvolto il Presidente di questa Camera, per il fatto che dobbiamo dare risposte anche in una direzione di tutela del tutela del principio di autodichia, che ci sia la necessità di mettere in campo immediatamente una Commissione monocamerale di inchiesta, avvalendoci delle misure previste dal nostro Regolamento e dalla strumentazione giuridica del Senato. Senato. Questa è la formula con la quale evitiamo colli di bottiglia, imbuti legislativi o rinvii e rimandi, e in tal modo diamo una risposta immediata di garanzia della tenuta e dalla salvaguardia delle istituzioni repubblicane.

Signor Presidente, innanzitutto, come Gruppo Lega, ci associamo alle parole che hanno espresso gli altri Gruppi, di solidarietà per l'attacco che avete subito lei e la sua famiglia.

un film che sembra del terrore. In procura nazionale antimafia ci sono stati 230.000 accessi abusivi in tre anni. Questo vuol dire che in procura nazionale antimafia, che dovrebbe essere la sede della sicurezza e della legalità, un accesso abusivo ogni minuto e ventuno secondi, e non è un caso che il partito più dossierato - come hanno detto tutti i giornalisti - sia stata la Lega: trovo che sia un attacco

Lega, dalla procura nazionale antimafia trovo che siano un qualcosa di inquietante, non solo per la Lega, ma per tutto il Parlamento e per la democrazia nel nostro Paese. Aggiungo che scinderei il problema in due categorie. Da un lato, c'è il tema della cybersicurezza, che riguarda le banche, le aziende e la politica; e su questo ci dobbiamo interrogare. Dall'altro, chi sono i mandanti? E con quali motivazioni stanno portando avanti un attacco alla democrazia? Su questo dobbiamo andare avanti, senza se e senza ma, negli interessi non solo della Lega, ma anche della democrazia del nostro Paese.

solidarietà per essere, statisticamente, il soggetto più coinvolto in qualsiasi dossieraggio. Del resto, è la seconda carica dello Stato e, dovendo rispettare la prima, per ragioni evidenti di garbo, cominciano dalla seconda, evidentemente proseguendo verso le altre.

senatore Boccia che invocava le dimissioni di questo o di quello. Noi abbiamo chiesto l'astensione di chi, essendo Vice Presidente dell'antimafia, non può indagare sulla sua attività precedente di procuratore nazionale antimafia. *(Applausi).* Infatti, in quanto a dimissioni e a incompatibilità, se vogliamo aprire un dibattito qui, lo apriamo, ma lo stiamo facendo già altrove. C'è la vicenda della banca di Bisceglie. Che un banchiere, non un bancario, entri in tutti i conti correnti è sorprendente, ed anche lì, signor Presidente, Ci sono norme che consentono di multare con cifre non irrilevanti le banche che commettono siffatti errori e io mi auguro che qualcuno cominci a punire.

vada avanti senza conflitti d'interesse interni, perché qui abbiamo quelli che fanno le domande e si danno le risposte; poi, quando ci sono intercettazioni di alcuni, non bisogna parlarne; prima, però, venivano pubblicate a puntate le intercettazioni degli altri.

funzioni bene. Abbiamo mille apparati, mille autorità e un milione di intercettazioni. Qualcosa non va e il Parlamento se ne deve occupare. Il mondo del centrodestra è statisticamente la vittima principale. E altri hanno al loro interno conflitti per cui stavano alla guida delle procure e devono indagare su se stessi. Noi tutto questo non lo possiamo accettare, dunque chiediamo trasparenza e discussione in Parlamento.

legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, in ordine alla documentazione fatta pervenire dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma, con riferimento all'acquisizione di corrispondenza del dottor Gennaro Sangiuliano,

preliminarmente, come lei sa, faccio presente che il sottoscritto è stato incaricato dalla Giunta di riferire oralmente all'Assemblea, così così come prescritto dall'articolo 135-*bis* del Regolamento del Senato, per quanto concerne la richiesta di autorizzazione *ad acta* di cui all'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989. A tale proposito si rappresenta che, in data 11 ottobre 2024, al Senato della Repubblica è stata notificata la richiesta di autorizzazione ad acquisire la corrispondenza dell'ex ministro della cultura Gennaro Sangiuliano da parte del collegio per i reati ministeriali del Tribunale di Roma e, in pari data, tale richiesta è stata trasmessa alla Giunta. La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 16, del 22 e del 29 ottobre 2024. L'istanza in oggetto si iscrive nell'ambito del procedimento pendente innanzi al predetto Tribunale dei Ministri presso il Tribunale di Roma a carico del dottor Sangiuliano per i reati di cui agli articoli 314-*bis* (indebita destinazione di denaro o cose mobili) e 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio) del codice penale, commessi in epoca anteriore al 5 settembre 2024, data della denuncia-querela presentata dall'onorevole Bonelli in relazione ad asserite irregolarità poste in essere dall'allora Ministro in ordine all'utilizzo di beni, servizi e mezzi dello Stato e di altri enti pubblici in favore di Maria Rosaria Boccia, nonché in ordine alla diffusione di informazioni riservate di origine ministeriale o governativa, che sarebbero state portate a conoscenza della stessa Boccia. L'autorità giudiziaria espone inoltre - come da notizie apprese da fonti aperte nell'ambito del successivo procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Roma, a seguito della denuncia presentata dal dottor Sangiuliano nei confronti della dottoressa Boccia risulta sia stato eseguito il sequestro di dispositivi elettronici e di telefoni cellulari da cui è stata estratta la copia forense dei documenti elettronici e delle comunicazioni intercorse anche con l'ex ministro. Il collegio dei reati ministeriali di Roma ritiene che tale documentazione informatica sia rilevante nel procedimento di cui trattasi, in ottemperanza alle conclusioni della Corte costituzionale, nella sentenza n. 170 del 2023 del 2023 sul conflitto di attribuzione sollevato per il caso del senatore Renzi. In virtù di tale sentenza, la Consulta ha stabilito che le comunicazioni mediante strumenti telematici come messaggi o posta elettronica siano da considerare corrispondenza e, come tale, soggetta per i parlamentari alle garanzie di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione; ha valutato che analoga autorizzazione vada richiesta per la corrispondenza dei Ministri, stante il disposto dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1989. In conclusione, il collegio procedente ha ritenuto che l'acquisizione e la successiva analisi della corrispondenza intercorsa tra la dottoressa Boccia e l'allora ministro Sangiuliano, già estratta dai dispositivi elettronici sequestrati all'indagata nel procedimento per reato comune, originato dalla denuncia dello stesso ex Ministro, sia possibile solo a seguito della concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 10 della citata legge costituzionale. Richiede quindi al Senato l'autorizzazione ad acquisire copia della copia forense integrale della memoria dei dispositivi sequestrati all'indagata e ad estrarre copia delle comunicazioni eventualmente intercorse con l'ex Ministro, che potrebbero essere utilizzate a fine di prova nel procedimento per i reati ministeriali innanzi descritti. Si fa presente che, in data 18 ottobre 2024, l'ex ministro Sangiuliano ha trasmesso alla Giunta una memoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto della richiesta del Tribunale dei Ministri, ritenendola inammissibile sul piano processuale e sostanziale. Occorre anche ricordare che l'articolo 10, primo comma, della citata legge costituzionale n. 1 del 1989 dispone che, nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonché gli altri inquisiti, che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, non possano essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione della corrispondenza, ovvero a perquisizioni personali e domiciliari, senza l'autorizzazione della Camera competente. Occorre considerare che la Giunta, nelle ipotesi di richieste di autorizzazione al sequestro di corrispondenza, deve valutare il *fumus persecutionis*. Tale *fumus* può rivestire una connotazione soggettiva, ossia riguardare un'inimicizia o un'intenzione persecutoria del magistrato procedente, e tale fattispecie viene connotata con l'espressione *fumus persecutionis* di primo grado. È tuttavia possibile che il *fumus* sia di secondo grado, cioè che lo stesso rivesta una connotazione oggettiva, legata alle modalità concrete con cui l'autorità giudiziaria ha proceduto. Sussiste poi un *fumus* di terzo grado, quando vengano ravvisati profili di illegittimità talmente macroscopici da radicare il sospetto di una persecutorietà. Nel caso di specie, non ci sono elementi per configurare il *fumus* di primo grado, né tantomeno profili di illegittimità tanto evidenti da consentire il radicarsi di un *fumus* di terzo grado. Sussistono invece profili idonei a configurare il *fumus* di secondo grado. Il carattere persecutorio dell'azione giudiziaria, sotto il profilo del *fumus* di secondo grado, può evincersi dall'assenza di un nesso specifico e motivato tra l'adozione del mezzo di ricerca della prova prescelto e la configurazione dei reati contestati, cosicché la generalizzata acquisizione del materiale probatorio, specie se telematico o telefonico, fa assumere al vincolo cautelare reale carattere esplorativo e sproporzionato (Cassazione penale, sentenza n. 11835 del 2022; anche, nella stessa vicenda, Cassazione penale n. 30225 del 2020), connotando il sequestro come onnivoro ed invasivo di una serie indifferenziata di dati personali (Cassazione penale 34265 del 2020 sullo stesso caso). Come nel richiamato precedente a cui si riferiscono le predette sentenze, anche nel caso di specie non è espressa la finalità probatoria del sequestro rispetto alla configurazione concreta dei reati perseguiti e l'indiscriminata acquisizione di una serie indefinita di dati, oltre che ledere la riservatezza dell'indagato, non appare finalizzata e funzionalmente correlata con la dimostrazione delle ipotesi di reato per cui si procede, manifestando anche in tal caso il carattere sproporzionato del provvedimento che fa radicare il plausibile sospetto della sussistenza del *fumus persecutionis* di secondo grado. Non è dato conoscere quali elementi stia ricercando l'autorità giudiziaria, né quali elementi indiziari siano finora emersi, né tantomeno quali siano eventualmente da verificare e provare. In altri termini, la genericità e la vaghezza delle finalità e delle motivazioni, nel caso di specie, lasciano emergere il *fumus persecutionis* di secondo grado. Si ricorda che il *fumus* non richiede una *probatio* della persecutorietà, ma solo la parvenza (il *fumus*, appunto) della stessa. Tutto quanto considerato ed esposto, la Giunta ha pertanto deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea il diniego di autorizzazione all'acquisizione di corrispondenza del dottor Gennaro Sangiuliano, Ministro della cultura *pro tempore*. Per mere esigenze di completezza istruttoria, *ad abundantiam,* si sottolinea infine che un altro aspetto problematico concerne la circostanza che le conversazioni e la corrispondenza telematica che riguardano l'ex Ministro sono già state estratte dai dispositivi elettronici e telefonici della dottoressa Boccia, indagata in un procedimento penale successivo rispetto a quello del dottor Sangiuliano e innescato su sua stessa denuncia. A tal proposito, occorre sottolineare che, pur non sottacendosi la giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di prerogative, che ha sempre affermato che tali norme sono di stretta interpretazione, in quanto derogano all'ordine generale della tutela giurisdizionale dei cittadini, tuttavia non può non evidenziarsi che all'epoca dell'acquisizione del materiale probatorio nel procedimento nei confronti della dottoressa Boccia era già fatto notorio che fosse pendente il procedimento penale per reati ministeriali nei confronti dell'ex ministro Sangiuliano. In un contesto di leale collaborazione tra poteri dello Stato, anche il giudice del procedimento per reato comune avrebbe dovuto porsi il problema della possibilità di estrarre tale corrispondenza senza la previa richiesta di autorizzazione, anche perché, diversamente opinando, sarebbe sempre possibile aggirare le prescrizioni della legge costituzionale n. 1 del 1989 attivando un procedimento penale a carico di uno stretto collaboratore di un Ministro ed acquisendo il materiale probatorio senza le limitazioni e le garanzie dell'articolo 10 della legge costituzionale, in elusione quindi del dettato normativo. Mi verrebbe da obiettare che, in tal caso, il procedimento per il reato comune era stato originato da una denuncia sporta dallo stesso ex Ministro, cui la garanzia del predetto articolo 10 si riferisce, in quanto, com'è noto, le prerogative e le guarentigie costituzionali a tutela del singolo, ma anche dell'istituzione rappresentata, non sono rinunciabili da parte dell'interessato. Gli elementi per ultimo citati potrebbero radicare un'invalidità per così dire derivata della stessa, essendo già stata estratta la corrispondenza in questione in un altro procedimento iniziato dopo quello per reato ministeriale. In altri termini, l'estrazione della corrispondenza in questione senza autorizzazione potrebbe inficiare in via derivata la legittimità della richiesta del Tribunale dei Ministri, che infatti chiede testualmente copia della copia, con tutti i risvolti di contraddizione sul piano logico, prima che giuridico. Se la copia è già stata estratta, la richiesta di copia della copia è illegittima, in quanto riveste una valenza in senso complessivo *ex post*, come fin qui spiegato, e non quindi *ex ante*, come sarebbe stato invece necessario. Si precisa infine che il Senato non ha alcuna conoscenza del contenuto di tutto il materiale acquisito dall'autorità giudiziaria ordinaria. In ogni caso, laddove fosse emersa una fattispecie di reato ministeriale, la procura avrebbe dovuto trasmettere d'ufficio la notizia di reato al Tribunale dei Ministri (che in fondo è quello che il Tribunale dei Ministri sta chiedendo a noi). Presenta profili anomali la *translatio probationis* avvenuta, nel caso di specie, da un processo a un altro di un mezzo di prova già formato e compiutamente acquisito in altro procedimento, senza che sia stata richiesta preventivamente l'autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro. Su questo tema ci siamo posti il problema di precedenti che non esistono nel nostro ramo del Parlamento; esistono invece precedenti alla Camera dei deputati. È chiaro che anche il fatto che vi siano precedenti o meno è questione valutativa da parte di ciascuno di noi, ma si richiama a tal proposito il precedente della Camera dei deputati del 2 febbraio del 1994, relativo al deputato Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica *pro tempore*, nonché il precedente, sempre della Camera dei deputati, del 5 agosto 1993 inerente al deputato Prandini nella sua veste di Ministro dei lavori pubblici *pro tempore.* In entrambi i casi predetti, l'autorizzazione a procedere fu presentata dall'autorità giudiziaria contestualmente alla richiesta di autorizzazione *ad acta*, con la conseguenza che in Assemblea, alla Camera dei deputati, si votò prima l'autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989 e solo successivamente l'autorizzazione *ad acta*, di cui all'articolo 10 della predetta legge costituzionale. Nel caso del ministro Sangiuliano, l'anomalia va ravvisata nella circostanza che è pervenuta in Senato esclusivamente la richiesta di autorizzazione *ad acta* e ciò nonostante la *traslatio* *probationis* cui si accennava in precedenza.

purtroppo ha perso la sua giovane e bella vita. A lei e ai suoi familiari va il cordoglio di tutto il Senato.

intervengo per dichiarare il voto contrario del Gruppo Italia Viva sulla relazione del senatore Paroli. Ci siamo avvicinati a questo caso con grande attenzione e grande cautela, grande cautela, dato che per molti versi costituisce un primo caso nella materia. Per esempio, abbiamo due procedimenti penali che stanno procedendo in parallelo e, come diceva giustamente il collega Paroli, in uno dei due, quello avviato dall'ex ministro Sangiuliano, la corrispondenza - di cui oggi il Tribunale dei Ministri chiede l'acquisizione - è già stata acquisita dalla Procura, per cui ci troviamo davanti a una richiesta della copia della copia forense di questa corrispondenza. Come dicevo, non è soltanto una questione di novità, ma anche di delicatezza del caso; da questi scranni, quando si parla delle prerogative parlamentari e della separazione dei poteri delle più alte cariche dello Stato, siamo particolarmente accurati nel valutarne la fondatezza e nel proteggerne l'esistenza, perché le riteniamo elementi preziosi nel bilanciamento dei poteri e del funzionamento della nostra Repubblica. Per quale motivo, allora, voteremo contro la relazione del collega Paroli? Il collega Paroli, come abbiamo appena sentito, ci dice che il Tribunale dei Ministri ha rilevato come rilevanti queste conversazioni, egli ritiene che invece si tratti sostanzialmente di una sorta di pesca a strascico. In sostanza, sulla base di un'ipotesi di reato molto fumosa, si chiede di ottenere le conversazioni per andare a trovare il reato; questo fa configurare una forma di *fumus persecutionis* e, di conseguenza, dovremmo rispondere negativamente al Tribunale dei Ministri. Sempre il relatore,

le conversazioni in vista della richiesta dell'autorizzazione a procedere. I due argomenti del collega non resistono, a mio

una pesca a strascico se, come dice il relatore, ci trovassimo in una situazione fumosa nella quale il reato non è chiaro. In realtà il Tribunale dei Ministri, quando si rivolge alla Giunta del Senato e al Senato, non parla di una rilevanza di queste conversazioni ai fini dell'indagine, ma le definisce indispensabili. La differenza - e la ragione della differenza - tra "rilevanti" e "indispensabili" è che queste conversazioni servono a verificare l'esistenza di un'ipotesi di reato molto specifica, che è quella dell'articolo 326 del codice penale, cioè della rivelazione di segreto d'ufficio.

qualsiasi reato di altro genere, come avverrebbe se volessi leggere per vedere se colui che ritengo essere il reo abbia per esempio scritto nelle *chat* di avere effettuato la malversazione, la concussione, la corruzione o quello che è. ci chiede come indispensabili quelle *chat* perché, nella rivelazione del segreto d'ufficio, la *chat* è il fatto criminoso. il fatto criminoso. Il crimine cioè non è provato attraverso la *chat*, ma è commesso attraverso di essa.

Questa differenza, secondo me, ci spinge a dire che il Tribunale dei Ministri si è ben comportato anche per ciò che attiene al secondo aspetto. Il Tribunale dei Ministri ci chiede subito di rinviare a giudizio l'ex ministro Sangiuliano? No, aver bisogno di vedere quegli atti per stabilire se il reato sia stato commesso e dunque, a quel punto, chiedere eventualmente l'autorizzazione a procedere,

chiedendo eventualmente il rinvio a giudizio. Badate bene, però, che il tribunale potrebbe anche decidere l'archiviazione, una volta lette quelle *chat*. La consegna delle *chat* paradossalmente - anzi, neanche paradossalmente - può essere determinata anche a favore della persona imputata del reato. Il Tribunale dei Ministri infatti potrebbe leggerle e non ravvedere alcuna fuga di notizie o rivelazione di segreto d'ufficio. Infatti, quando poi il Tribunale dei Ministri eventualmente dovesse chiederci di rinviare a giudizio l'ex ministro Sangiuliano, noi avremmo sessanta giorni, un tempo assai più lungo. La differenza dei termini, signor Presidente, ci spiega che i due atti sono di per sé indipendenti e non sono connessi. I precedenti cui si riferiva il collega Paroli, che riguardavano la Camera dei deputati, avevano a che fare con reati di tipo corruttivo e con fatti che erano esterni, quindi gli atti di cui si chiedeva l'acquisizione non erano

ministro Sangiuliano. Tra l'altro, voglio sottolineare che qui ci stiamo occupando di un reato ministeriale, perché l'ex ministro Sangiuliano non è un parlamentare. I casi nei quali sono state intercettazioni nei confronti di parlamentari sono differenti, perché il parlamentare è coperto a trecentosessanta gradi, data la propria funzione, mentre i membri di Governo, i Ministri in particolare, sono coperti da una legge costituzionale apposita, quando commettono reati nella loro qualità di Ministri, quindi cogliamo anche questa differenza. Per tutte queste ragioni, ritengo che la relazione del collega Paroli non sia condivisibile dal punto di vista tecnico: penso dunque che sia opportuno rispondere alla domanda del Tribunale dei del Tribunale dei Ministri, affinché si concluda l'attività istruttoria e poi il Parlamento possa decidere, nella sua amplissima autonomia, se vi saranno se vi saranno elementi sufficienti per il rinvio a giudizio oppure no. In questa fase preliminare, io direi che la richiesta del Tribunale dei Ministri è equilibrata equilibrata e accoglibile e tiene conto della più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, quindi della natura di corrispondenza anche delle *chat* di messaggistica immediata. Di conseguenza, il Gruppo Italia Viva-Il Centro-Renew Europe voterà contro la relazione che abbiamo appena ascoltato. Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, relativamente al caso di specie si è discusso in ogni dove nel globo terracqueo; finalmente, abbiamo l'opportunità di affrontare la questione nel luogo ad esso deputato. L'Assemblea è chiamata a decidere in merito alla richiesta di autorizzazione ad acquisire la corrispondenza dell'ex ministro della cultura Gennaro Sangiuliano da parte del Collegio per i reati ministeriali del Tribunale di Roma. I reati contestati sono: indebita destinazione di denaro o cose mobili e rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, in relazione ad asserite irregolarità poste in essere dall'allora Ministro in ordine all'utilizzo di beni, servizi e mezzi dello Stato e di enti pubblici in favore della dottoressa Boccia, nonché in ordine alla diffusione di informazioni riservate di origine ministeriale o governativa, che sarebbero state portate a conoscenza della stessa Boccia. A completamento della narrazione, si segnala che l'autorità giudiziaria, specificatamente il Tribunale di Roma, ha incardinato un procedimento che vede la suddetta in qualità di indagata per violenza o minaccia a corpo politico e lesioni, in seguito alla denuncia effettuata proprio dall'ex Ministro, dalla quale è scaturito il sequestro di dispositivi elettronici e di telefoni cellulari, da cui è stata estratta copia forense. Tutti i fatti sovraesposti sono di dominio pubblico, in quanto sono stati proprio gli stessi interpreti a monopolizzare l'attenzione mediatica sulla vicenda, mediante comparsate in *post* sui *social*, articoli di stampa e perfino utilizzando in maniera alquanto discutibile il telegiornale della rete ammiraglia della televisione pubblica, andando a creare una sovrapposizione quasi perfetta tra il TG1 e la *soap* «Un posto al sole». *(Applausi)*. Di lì a poco, le sacrosante dimissioni e l'avvicendamento con il quasi dottor Giuli. Dal posto al sole al pensiero solare è stato un attimo; sicuramente, uno spettacolo non edificante per la classe politica. La relazione conclusiva del relatore fa propendere l'Assemblea per respingere la richiesta di autorizzazione al sequestro di corrispondenza, in quanto sussistente il *fumus persecutionis* di secondo grado, legato alle modalità con le quali l'autorità giudiziaria ha proceduto. Intanto sorge spontanea una domanda: come può sussistere la persecuzione, se nell'ambito dell'altro procedimento - in cui l'ex Ministro figura come querelante - sono stati già sequestrati all'indagata Boccia i dispositivi dai quali sono state già estratte le comunicazioni ritenute rilevanti ai fini del reato per il quale si procede? Sussiste quindi sempre persecuzione quando un Ministro viene indagato, mentre non c'è mai quando il Ministro denuncia? Da ciò consegue che, relativamente a un procedimento in cui l'ex Ministro risulta il soggetto che ha sporto querela, egli può beneficiare di tutti gli strumenti investigativi di cui risulta dotato il codice, mentre nei casi in cui trattasi di reati ministeriali sussiste l'impedimento generato dal Può mai essere che un soggetto si trinceri dietro prerogative ministeriali e, al contempo, promuova un'azione penale sfruttando quegli stessi mezzi che all'altra parte sono preclusi, a causa del diniego all'autorizzazione, in ragione della forza dei numeri di maggioranza? È mai possibile che un soggetto venga eventualmente condannato per un reato comune sulla base del materiale estratto da un dispositivo, mentre - per un reato ministeriale che nulla ha a che vedere con la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo - quello stesso materiale sia impossibile da acquisire in ragione di una valutazione politica da parte del Senato? Così dispone l'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1989. La richiesta però dev'essere oggetto di un attento scrutinio da parte della Giunta e poi dell'Assemblea e può essere autorizzata non rigettata a prescindere. Il *fumus*, infatti, dev'essere riscontrato e nel caso di specie non lo si ravvede. L'integrazione di materiale istruttorio sarebbe stata necessaria ai fini della decisione in merito all'eventuale *fumus* anche in ragione del fatto che l'unico atto acquisito dalla Giunta è stata la memoria scritta dai legali, che hanno addirittura paventato, forse trascurando quanto disposto dalla legge costituzionale, anche l'illegittimità dell'acquisizione del materiale probatorio derivante dal sequestro del dispositivo mobile dell'addetto della dottoressa Boccia, in quanto manchevole della preventiva autorizzazione da parte del Senato. Il relatore, nella relazione conclusiva, parla di sequestro a carattere esplorativo e sproporzionato, onnivoro e invasivo di una serie indifferenziata di dati personali. dati personali. Quali sono gli elementi individuati dallo stesso al fine di motivare tale assunto ed esplicativi dell'abnormità della richiesta? Secondo lo schema dettato, la richiesta dell'autorità giudiziaria andrebbe rigettato in quanto in violazione della *privacy* dell'ex Ministro *privacy* dell'ex Ministro). Colleghi, è stato però proprio il dottor Sangiuliano a rendere edotta l'intera Nazione dei dettagli delle stesse conversazioni in quei diciassette minuti in cui ha strumentalizzato il più importante TG della RAI per autoassolversi, salvo poi dimettersi. Grazie, signor Presidente. Si fa riferimento anche a una scarsa motivazione nella richiesta da parte del Tribunale dei Ministri… PRESIDENTE. Parlava della Lazio, lo so.

quindi corretto monopolizzare il servizio pubblico d'informazione per autoassolversi senza contraddittorio; è giusto usufruire di tutti i mezzi quando l'esponente politico di appartenenza sia il querelante in un procedimento penale, mentre nei casi in cui trattasi di indagato si è pronti a raggiungere anche l'undicesimo livello di *fumus*, pur di sviare qualsiasi tipo di procedimento. Per le ragioni esposte, la richiesta del relatore dev'essere letta in chiave quasi provocatoria. A proposito di chiave, signor ex Ministro, *ma addo' sta a' chiave*? La chiave dov'è? *Cadeaux* vari. Per queste ragioni, dichiaro il voto contrario del Gruppo MoVimento 5 Stelle alla relazione conclusiva del relatore.

Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare il voto contrario dell'Alleanza Verdi e Sinistra sulla relazione della Giunta. Diversamente dalla maggioranza, infatti, riteniamo che questo caso specifico si discosti, e non poco, dai precedenti citati nella relazione, i quali si riferiscono a ipotesi di reato completamente diverse da quelle ipotizzate a carico dell'allora ministro Sangiuliano. Pensiamo infatti che in questo caso specifico il contemperamento degli interessi e dei diritti in gioco penda a favore dell'interesse pubblico alla conoscenza precisa dei fatti. La gravità di quanto accaduto, la risonanza mediatica data alla vicenda, ma anche e soprattutto sue possibili ripercussioni impongono, a nostro avviso, signor Presidente, che la magistratura sia autorizzata all'acquisizione dei dati necessari per appurare se, quando era Ministro, il dottor Sangiuliano abbia impiegato meno soldi pubblici per fini personali e per fare piena chiarezza sulla nomina di Maria Rosaria Boccia come consigliera del Ministro della cultura. Inoltre, diversamente da quanto ritenuto nella relazione, l'esposto a firma dell'onorevole Bonelli è sufficientemente circostanziato: si riferisce a ipotesi di reato specifiche ed è ampiamente documentato. Per questi motivi, signor Presidente, come anticipato, dichiaro il voto contrario dell'Alleanza Verdi e Sinistra

così similari, tanto da imporre - come ci hanno imposto la Giunta e così quest'Assemblea - di prendere una decisione che può anche segnare quasi un precedente nella casistica.

che, nei procedimenti per reati ministeriali nei confronti, in questo caso, di Ministri, non possano essere fatte intercettazioni, né sequestri, né si possa violare la corrispondenza, se non previa autorizzazione della Camera

dell'utilizzabilità di questo tipo di conversazioni, delle intercettazioni, come dell'utilizzo della corrispondenza, come nel caso di specie, seguono un principio, quello della valutazione fatta dalla Giunta se esista o meno il *fumus persecutionis*. Proprio nell'istanza che è stata portata avanti dal Tribunale dei Ministri si dice che questa documentazione si intende non solo importante, ma rilevante, anzi, indispensabile. Questo a dire che, per radicare il procedimento e costruire un'azione penale, è necessaria questa documentazione. Il magistrato del Tribunale dei Ministri non può conoscere il contenuto di questa *chat*, perché non è prodotta ancora in quel processo, quindi significa che ne ha una notizia. Da ciò, il fatto di volerla utilizzare a tutti i costi denota un intento chiaramente esplorativo per vedere se esista il reato.

abbiamo alcuni principi e passaggi logici: innanzitutto, com'è noto, almeno per ora nel nostro Paese vige l'obbligatorietà dell'azione penale, che subisce un'eccezione

del Ministro o della Ministra in questione, una doppia garanzia, perché prima di chiedere l'autorizzazione a procedere, cioè a svolgere un processo, che poi eventualmente sfocia nelle aule giudiziarie vere e proprie, debbono debbono essere svolte delle indagini, come riportato testualmente - non poteva essere diversamente - nella relazione del collega Paroli

archiviando, non si chiede neanche l'autorizzazione a procedere, a salvaguardia di chi ricopre l'incarico ministeriale. Siamo esattamente in questo caso. La questione sollevata è interessante:

tra i poteri dello Stato. Dico subito che le analogie con i precedenti, per usare un linguaggio processuale, non sono citazione in termini, nel senso che riguardano casi non paragonabili. Uno dei due era deciso contestualmente, perché c'era anche la richiesta d'arresto. Ora qui, in realtà, a garanzia del Ministro, prima di procedere oltre, si richiede di fare questa valutazione. Diciamo subito che l'argomentazione della relazione giunge a considerare di non concedere l'autorizzazione all'acquisizione di questi elementi di prova sotto il profilo del *fumus* cosiddetto di secondo grado: esso viene enucleato nei seguenti termini, cioè ci dev'essere un'assenza di nesso specifico e motivato tra l'adozione del mezzo di ricerca della prova prescelto e la configurazione dei reati contestati, quindi occorre assenza di nesso specifico e motivato. Non basta dire che sembra che ci sia un intento persecutorio:

un esposto che la richiesta del Tribunale dei Ministri - arrivata a noi - descrive nel senso che ci sono asserite irregolarità, poste in essere dal Ministro in ordine all'utilizzo di beni, servizi e/o mezzi dello Stato o altri enti pubblici in favore della signora Boccia e/o alla diffusione di informazioni riservate di origine ministeriale o governativa portandole a conoscenza della medesima. Questo è il richiamo all'esposto, seppur molto sintetico, ma che non può che ritenersi circostanziato,

una maggioranza della Giunta ci ha negato l'acquisizione di questo documento, pur richiamato nella richiesta del Tribunale dei Ministri, il quale pure aveva detto

nell'esposto, così com'è stato richiamato dalla relazione del Tribunale dei Ministri, il segreto d'ufficio richiede di per sé di acquisire la corrispondenza, perché è esattamente quello in cui si concreta: è il fatto, il corpo di reato e il mezzo. mezzo. Tra l'altro, è stata posta un'altra questione, *incidenter tantum*, sulla questione della non autorizzazione richiesta nel procedimento parallelo. qui l'estensione della garanzia del fatto che dev'essere chiesta l'autorizzazione anche per acquisire la corrispondenza fatta ai Ministri è esattamente nel perimetro dei reati ministeriali. L'altro procedimento è nato non per un reato ministeriale (non è tanto il problema della persona offesa o non offesa); certo, è una singolarità, ma ci chiederemo poi in futuro se questi casi possano essere affrontati diversamente; dal punto di vista strettamente formale però è diverso, mentre il parlamentare, anche se persona offesa e per qualsiasi reato, gode ovunque di tale garanzia. garanzia. In conclusione, stiamo parlando di un elemento di prova indispensabile e rilevante, che viene chiesto sulla base di un esposto che viene descritto come circostanziato, richiamando una descrizione di condotta, perché quando si dice

collegamento con questo fatto. Il nesso allora c'è, è dichiarato, è chiaro ed è motivato. Ci si richiama all'esposto sulle asserite irregolarità, pertanto è evidente che sussistano tutti gli elementi per non negare l'autorizzazione all'acquisizione di questo elemento di prova. Credo che sia giusto che ci interroghiamo,

palesare un andare a cercare a prescindere dalla sussistenza di un reato, per le funzioni che ha il Governo e per la separazione tra i poteri dello Stato. Ce lo siamo posti con grande serietà; però con altrettanta serietà, se vogliamo

Signor Presidente, onorevoli colleghi, in tutte le vicende procedurali che la Giunta per le immunità parlamentari rassegna all'Assemblea, inevitabilmente si intrecciano sullo sfondo pubblico e privato, a volte reati e peccati, vizi e virtù, errori ed espiazioni. È proprio per questo motivo però che l'Assemblea, con un voto politico, è onerata della necessità e della responsabilità di lasciare sullo sfondo e confinare in un angolo il voyeurismo d'accatto, l'informazione deformata e deformante di giornalismo di terz'ordine

a termini eterni e superiori come dignità, rispetto, reputazione, disciplina e onore. *(Applausi)*. Nel nostro dettato costituzionale è specificamente indicato che tutti i cittadini devono osservare lealmente la fedeltà alla Repubblica, alla Costituzione e alle leggi, però è anche indicato che i cittadini investiti di pubbliche funzioni hanno il dovere non soltanto di adempiervi, ma anche di farlo con disciplina e onore. Badate che la disciplina e l'onore sono termini che, mai come in questo caso, riportano alla mente anche fatti storici. Francesco I di Francia disse: tutto è perduto, fuorché l'onore. Egli fu accusato di dissolutezza. Re di Francia, uomo di cultura, mecenate delle arti, uomo del Rinascimento francese, che aveva portato Leonardo da Vinci alla sua corte, commise un unico, imperdonabile errore: quando ci fu il conflitto contro Carlo di Spagna, schierò in prima linea la sua cavalleria pesante, perché secondo gli schemi medievali quello era il sistema per vincere con gloria e onore; però l'errore di non poter utilizzare l'artiglieria contro il nemico, perché in quel momento per lui l'onore veniva prima di qualunque altra questione. la reputazione è ciò che gli altri pensano di noi; l'onore è quello che ciascuno di noi conosce di se stesso. La prima riflessione che s'impone dinanzi alla questione del ministro Sangiuliano che, a fronte dell'aggressione cinica, spietata, immorale e volgare contro la reputazione dell'uomo Sangiuliano, vi è più forte l'onore del Sangiuliano ministro. In secondo luogo, l'Assemblea è oggi chiamata non soltanto a una riflessione tecnica, ma anche a un voto di coscienza politica e cultura istituzionale. infatti valutare se e in che misura siano state rispettate le garanzie costituzionali, perché è questo che delinea l'architettura costituzionale di uno Stato di diritto. Intorno al tema delle immunità funzionali, che valgono tanto per i membri del Parlamento, quanto per i Ministri della Repubblica, si intreccia il nodo focale della separazione dei poteri e del loro equilibrio.

senza che vi sia l'autorizzazione della Camera competente, che in questo caso è il Senato della Repubblica. Questa norma costituzionale è servita proprio a riportare i reati ministeriali, che prima erano deferiti alla Corte costituzionale, nell'alveo del processo penale ordinario, ma con un filtro essenziale, quello politico dell'Assemblea parlamentare. È chiaro che era ed è necessario che il concetto della parità davanti alla giurisdizione, che è anche un corollario del principio di eguaglianza, va bilanciato con la garanzia della funzione di Governo. quindi oggi non può creare precedenti, non può ammettere che vengano svolte indagini preliminari senza che prima sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere. *(Applausi)*.

sulla base di un esposto generico, infondato, basato su fonti aperte e prodotto da un parlamentare dell'opposizione? Questa è la verità. è la verità. In questo momento, allora, se la Giunta è il luogo della riflessione tecnica, l'Aula è il luogo della decisione politica, per cui noi voteremo a favore della proposta del relatore contro la richiesta di acquisizione dei tabulati, perché - torno all'origine - il ministro Sangiuliano mai come in questo caso ha dimostrato nei fatti cosa significhi adempiere alle funzioni pubbliche con disciplina e onore. Appena si è palesato, anche solo per ipotesi, che vi fosse un conflitto d'interessi, egli non ha esitato un istante a difendere la ragione di Stato, giungendo persino a dimettersi e assumendosi responsabilità che non aveva, perché questo significa cultura politica per la destra: senso dello Stato, dirittura morale, rispetto delle istituzioni. *(Applausi)*. e rispetto alle vostre illazioni opponiamo la nostra sovrana indifferenza. l'uomo Sangiuliano, così pulito, capace e onesto, non va insolentito, ma rispettato. Il ministro Sangiuliano non va né perseguito, ma piuttosto ringraziato per quello che ha fatto non per il Governo, ma per la comunità nazionale, in un'operazione straordinaria di rilancio e valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Siamo convinti che anche il ministro Giuli andrà nella stessa direzione di difesa ad oltranza della nostra cultura nazionale, perché questo è quello che conta per un popolo che ha memoria ed identità e continuerà ad agire in discontinuità rispetto agli sconci del passato e in continuità, invece, con l'attività amministrativa e di governo che in due anni ci ha consentito di cambiare l'Italia. *(Applausi)*. È morto il re, viva il re!

e delle immunità parlamentari di negare l'autorizzazione all'acquisizione di corrispondenza del dottor Gennaro Sangiuliano, Ministro della cultura *pro tempore*, in ordine alla documentazione fatta pervenire dal collegio per i reati

senatore all'epoca dei fatti*** per consentire il procedimento parlamentare sulla questione dell'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole De Bonis, in attuazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

abnorme. Capita di tanto in tanto che la magistratura e le procure procedano nei confronti di parlamentari senza prima chiedere alla Giunta delle Camere di appartenenza una valutazione sull'insindacabilità *ex* articolo 68, ma in questo caso è successo che il tribunale è arrivato addirittura ad emettere sentenza di condanna nei confronti dell'ex parlamentare senza

della funzione del potere legislativo da parte del potere giudiziario. Se c'è quindi un caso nel quale il conflitto di attribuzione è

un caso nel quale, diversamente da com'è prescritto da una legge costituzionale, nonostante sia stata sollevata l'eccezione di sindacabilità dal parlamentare, il tribunale poteva negarla, ma aveva il dovere di trasmettere la copia degli atti al Senato, affinché questo si pronunciasse. Aveva due doveri: trasmettere e sospendere. Ciò invece non è stato fatto, nonostante le reiterate richieste,

Nella legittima separazione dei poteri e delle attribuzioni, il tribunale non si può sostituire a questa Camera. con grande tranquillità, perché sappiamo viceversa che, in altre situazioni, neanche questa Camera può sostituirsi o sovrapporsi alle spettanze della magistratura.

facciamo un lavoro molto accurato. Studiamo le carte, consapevoli della natura paragiurisdizionale dell'organismo del quale siamo parte e anche della delicatezza delle decisioni che prendiamo, perché si tratta della libertà personale e della fedina penale

e la magistratura davanti alla Corte costituzionale. Può essere un argomento molto tecnico, che magari non interessa alla maggior parte dei colleghi, ma, fino a quando l'Assemblea sarà sovrana e dovrà ratificare le decisioni della Giunta, credo che faccia parte dei nostri doveri d'ufficio dare a voi, colleghi, tutte le informazioni e spiegare il caso per come lo abbiamo

Li utilizzerò tutti, signora Presidente, o quanti deciderò di utilizzarne, avendo esaurito i miei argomenti. PRESIDENTE. Prego, senatore Scalfarotto. SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Noi abbiamo fatto anche in questo caso quello che si fa per valutare se l'articolo 68 sia applicabile, cioè se le opinioni che sono state espresse dal parlamentare siano state espresse nell'esercizio della medesima attività parlamentare.

ci ha spiegato che quello di cui si trattava era un caso di cui egli si era occupato ampiamente durante la sua attività parlamentare e in generale politica (ma in particolare in quella parlamentare). Verificato che questi presupposti, che sono quelli dettati dalla giurisprudenza costituzionale, fossero presenti, abbiamo quindi stabilito a maggioranza di sostenere la tesi della relatrice, che era quella di riconoscere l'insindacabilità *ex* articolo 68. Di conseguenza, in con questa posizione, il mio Gruppo voterà a favore dell'insindacabilità, quindi a favore della relazione della relatrice.

intervengo solo per annunciare il voto favorevole del Partito Democratico. Questo è un classico caso in cui le dichiarazioni del parlamentare sono state numerose e precedute da interventi in Aula, interrogazioni e finanche un impegno su una Commissione che si occupa specificatamente del tema.

rese dal senatore Carlo Calenda, oggetto del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma, non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni

e delle immunità parlamentari sono state già stampate e distribuite. Nei due casi di specie la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha deliberato, all'unanimità, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere con riguardo all'acquisizione dei dati di traffico telefonico/telematico in questione relativi ad utenze telefoniche in uso al senatore Claudio Lotito, ai sensi dell'articolo 68,

Presidente, desidero solo aggiungere che, nella seduta del 6 agosto 2024, il senatore Lotito si è presentato e ha ribadito egli stesso il consenso all'acquisizione dei dati. Avverto sin d'ora che, pur svolgendosi un'unica discussione, l'Assemblea delibererà separatamente su ciascuna delle proposte della Giunta.

che procede di aver seguito appunto questi passi. Abbiamo sentito il senatore Lotito, che è venuto personalmente in Giunta a dirci che autorizzava l'acquisizione degli atti. Ovviamente, come accade in tutti questi casi, non abbiamo alcuna ragione per votare contro e voteremo a favore.

per cui abbiamo votato favorevolmente in Giunta. Il perché era molto semplice. Il senatore Lotito ha chiesto che venissero trasmessi gli atti: quindi che cosa dire di più? Ne approfitto però per fare una riflessione proprio sull'articolo 68, nello specifico sul comma 3, che richiede l'autorizzazione del Parlamento per l'acquisizione di intercettazioni o dati comunicativi che riguardano i parlamentari. Questo articolo rappresenta una garanzia fondamentale non solo per la tutela delle prerogative parlamentari, ma anche per assicurare trasparenza e rigore nel bilanciamento tra esigenze - come diceva il collega Rastrelli - equilibrio tra esigenze investigative e rispetto delle funzioni istituzionali. L'articolo 68, nella sua applicazione, garantisce che qualsiasi richiesta da parte dell'autorità giudiziaria sia sottoposta al vaglio parlamentare giustissimo - assicurando così una più attenta e corretta analisi probatoria dei tribunali. Questo meccanismo permette di operare con maggiore trasparenza e responsabilità, evitando il rischio di abusi o scorrettezze che potrebbero compromettere non solo i singoli parlamentari, ma anche - e lo sottolineo - il corretto funzionamento delle nostre istituzioni democratiche. Nel caso specifico, voglio brevemente ringraziare il senatore Lotito per la sua cooperazione il suo consenso, espresso in modo diretto, trasparente e univoco. Egli ha dimostrato l'importanza di una collaborazione tra i poteri dello Stato, in un'ottica di rispetto reciproco È un esempio positivo di come l'applicazione dell'articolo 68 non debba essere vista come una protezione ad ogni costo, ma piuttosto come uno strumento per assicurare che la giustizia si muova sempre nel rispetto dei principi costituzionali. Mi spingo oltre. Secondo me, il gesto del senatore Lotito mostra più di quanto vorrebbe: non solo trasparenza di chi non teme, ma soprattutto le oscure ragioni di chi invece utilizza l'articolo 68

Signor Presidente, anticipiamo il voto a favore del Gruppo Lega, sottolineando come sia sottratto comunque alla disponibilità, anche da parte del senatore, l'utilizzo di questo tipo di dati del traffico

Signor Presidente, anche noi voteremo a favore della relazione per le ragioni che sono state già ben argomentate *in primis* dal senatore Scalfarotto. Si tratta di un procedimento in cui il senatore Lotito è persona offesa; lui stesso ha chiesto l'acquisizione dei tabulati e delle sue conversazioni per accertare i reati che ha denunciato, per cui non ci sono ragioni che ostano a concedere l'autorizzazione. Ovviamente si deve passare dal Senato perché è un diritto non rinunciabile, quello relativo alle prerogative del parlamentare, quindi si passa da questa sede, ma in questo caso ovviamente non ci sono ragioni ostative, per cui voteremo a favore. Questa dichiarazione di voto vale anche per il prossimo documento. simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione all'acquisizione dei dati di traffico telefonico/telematico, in sola entrata, delle utenze in uso al senatore Claudio Lotito, persona offesa dal reato e a cui tutela si procede, per il periodo di tempo compreso tra il mese di agosto 2023 e il giorno e il giorno dell'esecuzione del decreto di acquisizione, nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Roma. *(Segue la votazione)*. la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione all'acquisizione dei dati di traffico telefonico/telematico, in sola entrata, delle utenze in uso al senatore Claudio Lotito, persona offesa dal reato e a cui tutela si procede, per il periodo di tempo compreso tra il mese di aprile 2024 e il giorno dell'esecuzione del decreto di acquisizione, nell'ambito di un procedimento penale pendente dinanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario di Roma. *(Segue la votazione)*.

costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La relatrice, senatrice Cucchi, non intende intervenire.

la ex senatrice Iori ha correttamente azionato l'articolo 68, perché tale articolo è in Costituzione: quindi non c'è una correttezza

Il collega Lotito ha tanti pregi, ma in questo caso si è limitato a fare quello che gli serviva, cioè far partire la querela che egli stesso aveva presentato. Sarebbe stato che avesse fatto una querela e poi fosse venuto in Giunta per chiedere di non dire niente ai magistrati. Non c'è quindi una correttezza di chi utilizza l'articolo 68 e una scorrettezza da parte di chi non lo utilizza, fintanto che l'articolo 68 c'è, la collega Damante ha l'iniziativa legislativa, come tutti i parlamentari, quindi può presentare un bel disegno di legge di modifica dell'articolo 68, così eliminiamo l'insindacabilità dei voti e delle opinioni dei parlamentari. Finché c'è però, dato che parliamo tutti della bellezza della nostra Costituzione, o la Costituzione è bella tutta, o non può esserlo soltanto a pezzi. È bella anche quando protegge il Parlamento e consente ai parlamentari di svolgere la loro funzione, non di portavoce, ma di rappresentanti democraticamente eletti dal popolo in piena libertà e senza che vi siano azioni di disturbo che possano limitare quelle libertà. Detto questo, il caso della senatrice Iori è da manuale,

perché il Giarrusso era stato nominato coordinatore di un osservatorio sui concorsi universitari e molti avevano fatto notare che il suo *curriculum* non era assolutamente adeguato; tra questi vi era anche la senatrice Iori, che era stata anche cofirmataria di un'interrogazione su un caso politico: il Ministro che nomina come consulente una persona che non ha i titoli per essere nominata. Il Giarrusso ha querelato la Iori la Iori per diffamazione e la Giunta si è limitata a fare quello che deve fare, cioè a leggere l'articolo 68 e a verificarne l'applicabilità nel caso concreto. Cosa dice la Corte costituzionale? Se le opinioni Se le opinioni o i voti sono stati espressi da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni e quindi - dice la Consulta - sono rinvenibili anche in un atto parlamentare e sono contemporanei all'espressione che viene fatta fuori dal Parlamento, quell'opinione è insindacabile: ciò perché è l'espressione della libertà del rappresentante del popolo, che deve poter dire, per esempio, che un Ministro ha preso una decisione sbagliata. Abbiamo fatto quindi questa verifica: la relatrice Cucchi ha concluso dicendo che era proprio un caso di scuola, da manuale; voglio quindi annunciare il voto favorevole alla relazione della senatrice Cucchi, sottolineando anche che non stiamo concedendo un privilegio alla senatrice Iori. Abbiamo soltanto fatto in modo che quella persona, che rappresentava decine di migliaia di elettori che l'avevano portata qui, stava esprimendo una valutazione più che legittima nei confronti dell'autorità di Governo: quell'espressione, per definizione, non può essere dunque bloccata da un'azione giudiziaria, perché, se così fosse, tutti coloro che sono seduti in questo altissimo consesso non potrebbero portare a non potrebbero portare a termine e condurre correttamente le responsabilità per le quali sono stati mandati qui dentro. *(M5S)*. Signora Presidente, il Gruppo MoVimento 5 Stelle non concorda nella maniera più assoluta con le conclusioni proposte dalla relazione, individuate dalla relatrice. Mi devo allacciare anche a quello che ha detto il senatore Scalfarotto, che mi ha preceduto, perché, secondo la relatrice e anche secondo il Gruppo Italia Viva, non c'è nessuna discrasia e

non è così e c'è anche la motivazione, che non è solo tecnica, ma ci sarebbero anche altre considerazioni da fare. Intanto i fatti quali sono? Il 5 settembre 2018, su una testata giornalistica *online*, Iori, senatrice all'epoca dei fatti, etichettava l'allora segretario particolare del vice ministro all'istruzione, Dino Giarrusso, come venditore di bufale antiscientifiche e campione TV dell'antiscienza e dei processi TV, articolo intitolato «Dino Giarrusso? La competenza non è più una virtù»: questo il 5 settembre 2018. In data 11 settembre 2018, invece, veniva presentata al Senato un'interrogazione avente ad oggetto la vicenda commentata nel suo articolo: un'interrogazione sul tema presentata solo successivamente, proprio per giustificare, forse retroattivamente, dichiarazioni forti ed offensive. Aula siamo quindi stati chiamati a capire se tali manifestazioni verbali e comportamenti tenute dalla parlamentare siano assistite dalla prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Colleghi, vi chiedo: può mai la caratteristica dello *status* parlamentare essere estesa sino a ricomprendere anche gli insulti (di questo parliamo), solo perché non vengono giustificati come opinioni politiche? Siamo sicuri che questi insulti fossero opinioni politiche? Aggiungo che si arrogano anche il diritto di dire che

il cofirmatario non ha lo stesso potere del primo firmatario. L'unico che può disporre, modificare, ovvero decretare la morte dell'atto mediante il ritiro è proprio il primo firmatario; il cofirmatario ha una funzione meramente secondaria, tanto che, in caso di un'eventuale riformulazione dell'atto, non ha alcun potere di intervento, se non quello di chiamarsene fuori ritirando la firma. Inoltre, l'atto di sindacato ispettivo citato nella relazione è relazione è cofirmato da altri 25 senatori, colleghi di Gruppo. Sulla base dell'assunto che tale atto sia sufficiente a far dipendere la sussistenza dell'insindacabilità, se ne dedurrebbe che, qualora tutti e 26 i cofirmatari avessero posto in essere manifestazioni verbali e comportamenti materiali volti a denigrare il Giarrusso di turno, sarebbero comunque stati coperti dall'insindacabilità. Ciò risulta assolutamente in distonia rispetto alla *ratio* dell'istituto in parola. Questa interpretazione estesa dell'articolo 68 della Costituzione, che sembrerebbe offrire un'immunità collettiva ai membri di uno stesso Gruppo, appare costituzionalmente inappropriata. Diversi sono i pronunciamenti della Corte costituzionale che ribadiscono che una simile lettura dell'articolo 68 porterebbe a giustificare il comportamento di un parlamentare per atti *intra moenia* posti in essere da altri, perché semplicemente appartenenti allo stesso schieramento (sentenze n. 146 del 2005, n. 347 del 2004, n. 249 del 2006 e n. 97 del Questo significherebbe davvero oltrepassare i confini costituzionali. Vale la pena ricordare che l'immunità parlamentare prevista dall'articolo 68 della Costituzione fu pensata per impedire che la libertà dei parlamentari venisse limitata dalle autorità Era quindi un articolo di garanzia per il lavoro dei parlamentari e non una garanzia di impunità per i parlamentari. Usare l'immunità parlamentare per arrogarsi il diritto di insultare un cittadino o chicchessia vuol dire svilire l'importanza dell'istituto. dell'istituto. È una prassi che rischia di trasformare una prerogativa nata per tutelare la libertà di discussione in un inaccettabile privilegio di carattere personale. Non stupiamoci se poi i cittadini indicano l'immunità parlamentare tra i più odiosi privilegi della politica. L'ho detto e lo ripeto: impegniamoci affinché rimanga immunità parlamentare e non impunità parlamentare.

anche noi voteremo a favore della proposta della Giunta, perché ne condividiamo le motivazioni. Penso che questo sia un caso di scuola del funzionamento dell'articolo 68 della Costituzione, a tutela delle prerogative dei parlamentari.

siano state in qualche modo riprese e utilizzate anche in atti cosiddetti *intra moenia*, cioè dentro questo Palazzo. In questo caso, le dichiarazioni della nostra ex collega Vanna Iori hanno lo stesso identico contenuto di quella interrogazione depositata depositata pochi giorni dopo dalla stessa senatrice e quindi in uno stato di sostanziale contestualità temporale che è un requisito richiesto dalla Corte costituzionale. non riesco bene a comprendere gli argomenti che ho appena sentito, come quello per cui se un senatore firma insieme ad altri di fatto non firma, perché il firmatario sarebbe solo il primo e gli altri non contano nulla: se un senatore firma insieme ad altri senatori, ha firmato quell'atto e quindi ne assume totalmente totalmente la paternità. Pertanto, in questo caso mi pare che siamo esattamente nell'ambito di applicazione dell'articolo 68. Tra l'altro, nelle dichiarazioni della senatrice Iori dato riscontrare alcun insulto, quindi non siamo dentro quell'eccezione che è stata evocata, per cui francamente non trovo una ragione che sia una per negare in questo caso l'applicazione *de plano* dell'articolo 68 alle dichiarazioni

senatrice all'epoca dei fatti, oggetto del procedimento penale pendente presso il predetto Tribunale di Reggio Emilia, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. La relatrice, senatrice

Tribunale di Roma, non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

ha trasmesso al Senato, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140, copia degli atti relativi al procedimento penale n. 21941/2024 R.G.N.R. - n. 17589/2024 R.G. pendente nei confronti del senatore Carlo Calenda per accertare se le condotte oggetto del procedimento penale *de quo* integrino o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Tale procedimento ha ad oggetto il reato di diffamazione aggravata ed è originato da una querela sporta dall'onorevole Mario Clemente Mastella in relazione alle affermazioni pubblicate dal senatore Calenda in data 3 aprile 2024 sulle proprie pagine di profilo dei *social network* X (denominato in passato Twitter), Facebook e Instagram, contenute in un intervento in risposta al *post* pubblicato sul profilo Facebook dall'onorevole Emma Bonino. Le dichiarazioni a cui si riferisce la querela sono sostanzialmente le seguenti: «Non ha alcun senso portarsi dietro, sia pure per interposta persona, Cuffaro, Cesaro e Mastella. La cultura della mafia è l'opposto della cultura europea. Non ha alcun senso candidare in UE […] chi è pagato da dittatori stranieri. Chiamare la lista Stati Uniti d'Europa non può coprire personaggi e comportamenti che rappresentano l'opposto dei valori valori europei». L'onorevole Mastella aveva ritenuto tali espressioni lesive della propria reputazione, con particolare riguardo all'accostamento della sua persona e della sua storia politica alla mafia e a personaggi politici che sono stati coinvolti in vicende giudiziarie per fatti di mafia. Il senatore Calenda, nella memoria scritta depositata anche in sede di audizioni dinanzi alla Giunta, ha precisato che - come risulta da una nota diramata dal proprio partito lo stesso 3 aprile 2024 non aveva inteso definire «mafioso» l'onorevole Clemente Mastella, in quanto il riferimento alla cultura della mafia nelle dichiarazioni contestate atteneva esclusivamente alle vicende giudiziarie di Salvatore Cuffaro. Sotto altro profilo, ha sostenuto che, in ogni caso, le sue affermazioni rientrassero nel perimetro di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in virtù del nesso funzionale ribadito dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 104 del 2024. Alla luce di tali principi, a suo avviso, avrebbero dovuto soccorrere nel caso di specie gli interventi del deputato di azione Antonio D'Alessio, il quale, nelle date del 23 maggio, 11 giugno e 19 luglio 2024, aveva evidenziato l'importanza della lotta alla mafia e alla cultura mafiosa. Nel corso dell'esame dinanzi alla Giunta, richiamando la giurisprudenza costante della Consulta in materia di insindacabilità parlamentare, è stato rilevato che nel caso in esame non si è rinvenuto alcun atto parlamentare, né contestuale né immediatamente precedente o successivo, nel quale il senatore Calenda tratti la questione affrontata nelle dichiarazioni rese all'esterno delle Aule parlamentari. È stato peraltro rammentato che la stessa Corte costituzionale ha chiarito come la verifica del nesso funzionale tra dichiarazioni rese *extra moenia* ed attività tipicamente parlamentare, nonché il controllo sulla sostanziale corrispondenza tra le prime e le seconde, debbano essere effettuati con riferimento alla stessa persona, mentre sono irrilevanti gli atti di altri parlamentari, non potendosi configurare una sorta di insindacabilità di gruppo. Per tali motivi, nella seduta del 1° ottobre 2024 la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea l'insussistenza della insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Calenda nel procedimento *de quo*.

e lo stesso è il compito della Giunta, che opera verificando se le opinioni espresse dal parlamentare siano suscettibili di essere considerate insindacabili *ex* articolo 68. Nel caso precedente abbiamo visto che le parole incriminate, che avevano fatto sentire diffamato colui che aveva poi querelato la ex collega, erano state dette in sede politica e contenute

nel senso che qui abbiamo un *tweet* che ha fatto sentire una terza persona, in questo caso l'onorevole Mastella, colpito nella sua onorabilità. Dobbiamo quindi verificare se possiamo sacrificare il diritto del cittadino, che si è sentito leso

il senatore Calenda ha detto che non si riferiva all'onorevole Mastella e quindi non voleva offenderlo. Per questo ha esibito un'agenzia che diceva che fonti del suo partito interpretavano il suo pensiero, ma l'onorevole Mastella non ha ritirato la querela,

nei confronti dell'onorevole Mastella, come nel caso precedente nei confronti dell'onorevole Giarrusso, fosse contenuta in atti parlamentari. Purtroppo di questi atti parlamentari non vi è traccia.

L'onorevole Calenda ha detto che il suo partito è contro la mafia. Il problema è che l'articolo 68 non copre i segretari di partito, copre i parlamentari. Non si può cioè configurare l'insindacabilità *ex* articolo 68 se ad 68 se ad esprimersi in quel modo è stato un collega di partito, tanto più se sta in una Camera diversa da questa. Fondamentalmente a noi è mancato il collegamento, che deve esserci, tra le espressioni rivolte all'onorevole Mastella e un atto parlamentare, compiuto dal senatore Calenda in quanto parlamentare, che appunto dicesse qualcosa legato alla cultura della mafia e alla persona dell'onorevole Mastella. comprendendo che si tratta in questo caso di una critica politica, posto che la persona che si è sentita lesa permane nella sua convinzione - e posto che purtroppo non c'è un legame funzionale tra le cose dette in quel *tweet* e l'attività parlamentare del senatore Calenda (tant'è che ha dovuto ricorrere ad atti appartenenti ad altro parlamentare) - diventa complesso riconoscere l'esercizio di una prerogativa che appartiene ai parlamentari, di cui all'articolo 68 della Costituzione. pertanto aderito alle conclusioni della senatrice Lopreiato e voteremo a favore della relazione.

cosiddetti *intra moenia*, cioè tipici parlamentari, nei quali fossero riportate le stesse considerazioni che erano state fatte esternamente, così abbiamo dovuto procedere anche in questo caso a tale verifica, che però

ci sia una composizione delle ragioni di doglianza dell'onorevole Mastella nei confronti del senatore Calenda, perché si tratta evidentemente di una dichiarazione con la quale il senatore Calenda, come egli stesso ha ripetutamente detto, non intendeva assolutamente accostare il nome di Mastella alla criminalità organizzata. pertanto che ci siano tutti i presupposti perché questa vicenda non prosegua nelle aule di tribunale, ma, per quanto ci è dato decidere qui, non possiamo che votare a favore della relazione della relatrice. Signor Presidente, la relatrice, senatrice Lopreiato, ha messo bene in evidenza i tratti salienti di questa vicenda, ragion per cui non tornerò sui fatti che ha evidenziato. non convince fino in fondo, perché nasconde zone d'ombra legate a un giustizialismo superato dal tempo e sembra celare regolamenti di conti all'interno del campo largo (o campo Certamente le affermazioni del collega Calenda, nella lettura complessiva delle frasi pubblicate sui *social network*, risultano di portata lesiva per l'onorabilità del querelante, con particolare riguardo all'accostamento dell'onorevole Mastella alla cultura mafiosa o comunque a personaggi politici che sono stati coinvolti in vicende giudiziarie per fatti di mafia. Mi preme però sottolineare che, pur valutando positivamente alcuni passaggi della relazione, non posso negare le mie perplessità, condivise dal mio Gruppo, in riferimento alla differenza ivi nettamente tracciata tra attività politica e attività parlamentare. A nostro parere, non è possibile delineare una demarcazione netta tra i due aspetti, pur essendo indiscutibile che le guarentigie dei parlamentari vadano interpretate sempre all'interno della cornice tracciata dalla Costituzione e dalla Corte costituzionale. A tal proposito, ricordo come l'ordinamento costituzionale italiano abbia compiuto una scelta chiarissima: proteggere il parlamentare dal punto di vista funzionale laddove vi sia un nesso stretto e qualificato con l'attività parlamentare. Con la sentenza n. 104 del 2024, la Consulta ha però evidenziato come i parametri storicamente enucleati per individuare il nesso funzionale allo svolgimento dell'attività parlamentare siano meri indici rilevatori, non potendo costituire un limite al ruolo che la Giunta deve avere nell'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, alla fattispecie concreta. La Giunta deve pertanto rivendicare il ruolo di organo che detiene il potere di valutare, in modo responsabile, ma anche elastico, la delimitazione dell'area del nesso funzionale in senso costituzionalmente orientato. Proprio per questo il nostro Gruppo aveva chiesto alla relatrice di rivedere il percorso motivazionale, discostandosi dalla logica restrittiva che era posta a fondamento della sindacabilità in sede giurisdizionale delle affermazioni rese dal senatore Calenda. Il nostro ruolo oggi è decidere se l'opinione espressa dal senatore Calenda rientri nell'esercizio delle attività politico-parlamentari. Se, a parere del sottoscritto, è difficile immaginare il contrario, è altrettanto difficile esaminarla alla luce delle circostanze in cui si è delineata la fattispecie incriminatrice e soprattutto dei condizionamenti politici che hanno portato alla stesura della relazione finale. Per questi motivi, il Gruppo Fratelli d'Italia si asterrà. scrutinio simultaneo della proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di ritenere che le dichiarazioni rese dal senatore Carlo Calenda, oggetto del procedimento penale pendente presso il Tribunale di Roma, non costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e non ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione. *(Segue la votazione)*.

Comunico che in data 28 ottobre 2024 è stato trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento il seguente disegno di legge di iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia: «Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 2024, n. 158, recante disposizioni urgenti in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale» (1280), già presentato alla Camera dei deputati il 23 ottobre 2024.

Signor Presidente, il 25 ottobre dello scorso anno, alla soglia dei novantun anni, ci lasciava il professor Pietro Nervi, nato in Liguria e diventato trentino a pieno titolo, professore emerito dell'Università di Trento, dov'è stato titolare dei corsi di economia delle comunità europee e di economia montana e forestale. Per più di vent'anni è stato docente all'Istituto agrario di San Michele all'Adige, direttore della Scuola superiore di servizio sociale, vero e proprio inventore dell'Università della terza età e del tempo disponibile. Il professor Nervi ha insegnato ai suoi allievi il rispetto per la terra, ai giovani l'amore per lo studio e agli anziani che non si finisce mai di imparare, ma anche queste Aule gli devono tanto. Egli fu l'autore del testo di legge approvato in via definitiva dal Parlamento il 20 novembre 2017, la legge n. 168, sulle norme in materia di domini collettivi. Nervi è stato infatti uno dei padri nobili della tutela degli usi civici, cui ha dedicato studi e convegni, dibattiti e un impegno fuori dall'ordinario per far comprendere che le terre di antico godimento collettivo non potevano essere indirizzate a finalità diverse da quelle dell'interesse generale. Laureatosi nel 1957 in scienze agrarie, collaborò prima con una Commissione ministeriale chiamata a occuparsi dei problemi del settore agricolo. Poi, nel 1961, fu chiamato a Trento per contribuire alla stesura del Piano urbanistico provinciale, il primo piano urbanistico. A un anno dalla sua scomparsa vogliamo ricordarlo come colui che ha salvato il Trentino da chi vagheggiava una megalopoli lungo la Valle dell'Adige, una città lineare di 80 chilometri tra Bolzano e Rovereto. Pietro Nervi, invece, contribuì alla nascita dei comprensori, della città diffusa, in grado di frenare lo spopolamento delle valli con la delocalizzazione dei servizi. Un mese prima della scomparsa, il sindaco di Trento ha voluto attribuirgli la massima onorificenza della città, l'Aquila di San Venceslao, antico sigillo del Principato tridentino. La memoria del professor Pietro Nervi rende onore a uno degli ultimi costruttori di un Trentino autonomo, orgoglioso della propria storia e strenuo difensore della sua dimensione comunitaria. Per le future generazioni, un esempio fulgido di impegno intellettuale e civile, sempre a difesa del bene comune e dell'interesse generale. Signor Presidente, prendo la parola in quest'Aula, che è il tempio della democrazia, per denunciare un grave episodio di intolleranza politica avvenuto oggi stesso presso la facoltà di lettere dell'Università di Ferrara, la mia città. È successo infatti che, mentre uno studente di Azione Universitaria (che, come tutti sanno, è l'organizzazione dei giovani universitari vicina a Fratelli d'Italia) Fratelli d'Italia) stava illustrando il programma della propria lista in occasione delle prossime elezioni universitarie, si sia sentito apostrofare come fascista dalla stessa insegnante che si trovava seduta accanto a lui in cattedra, di fronte agli studenti che stavano in ascolto. Alla risposta del ragazzo, che non si interessava di politica, ma solo di rivendicazioni studentesche, l'insegnante replicava tuttavia, testualmente, che Azione Universitaria è fascista e che anche il Governo Meloni è fascista. Questo è un professore universitario nell'esercizio delle sue funzioni. Cari colleghi, è un brutto episodio, che purtroppo non fa onore all'Università di Ferrara e che mi auguro venga adeguatamente sanzionato, perché i giovani non hanno bisogno di cattivi maestri che abusano della propria posizione per diffondere odio tra le giovani generazioni, ma di credere nel valore del reciproco rispetto, sul quale sempre deve fondarsi il confronto, pur nella legittima diversità di opinioni. PRESIDENTE.

Si sta alimentando un clima di odio e di violenza che credo sia davvero un cattivo messaggio ai più giovani. È difficile riuscire a insegnare qualcosa di buono e una parola di pace o comunque di confronto civile, lasciando che queste cose si moltiplichino e che queste espressioni di odio e di intolleranza nei confronti degli avversari politici, magari perché c'è la campagna elettorale in corso, avvengano senza nessuna censura. Sentivo davvero il bisogno di